relatore*. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, lasciatemi ricordare le parole pronunciate dal presidente del Consiglio Matteo Renzi all'indomani della strage al Théâtre Bataclan di Parigi: «Reagiamo al terrorismo con più teatri e più cultura», un messaggio politico forte e inequivocabile, largamente condiviso dall'opinione pubblica e dalle forze politiche. La cultura, la musica, la danza, il teatro stimolano la libertà di espressione contro l'oscurantismo degli integralismi, rafforzano il senso di appartenenza ad una comunità, favoriscono la coesione sociale, l'integrazione e la condivisione di valori identitari. Per questo in quei giorni drammatici il Governo decise di stanziare un miliardo in sicurezza ed uno in cultura, perché l'Europa, scossa dall'orrore, potesse reagire

la discussione del disegno di legge Pagliari, raccogliendo l'unanime volontà della Commissione di contribuire al sostegno di due importanti Festival nazionali, il Festival Verdi e il Festival Romaeuropa, non soltanto per la loro valenza artistica, estetica e culturale, ma anche per quella morale, civile e sociale del Paese e dell'Europa intera. Il 2013 è stato l'anno del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi; egli è infatti nato a Le Roncole (oggi Roncole Verdi) frazione di Busseto, in provincia di Parma, il 10 ottobre 1813. Con la legge 12 novembre 2012, n. 206, il Parlamento ha voluto celebrare la figura del Maestro dichiarando il 2013 «anno verdiano», riconoscendo i luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della

della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi. Le celebrazioni per il bicentenario hanno richiamato a Parma, nei luoghi verdiani, in Italia e nel mondo una crescente attenzione alla figura del Maestro di Busseto; attenzione che desideriamo mantenere viva una volta terminate le celebrazioni, proprio perché il Maestro di Busseto e le sue opere rappresentano un valore fondamentale per l'identità nazionale. A questo fine, la presente proposta di legge intende riconoscere alla Fondazione Teatro Regio di Parma, per la realizzazione del Festival Verdi, un contributo annuale di importo pari a quello che che la legge 20 dicembre 2012, n. 238, ha riconosciuto ad altri festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. Il Festival Verdi nasce nella seconda metà degli anni Ottanta ed ha avuto luogo fino al 1993, per poi essere reintrodotto nel 2001 in occasione delle Celebrazioni nazionali del centenario verdiano. Il Festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma, capace di estendere l'attività produttiva anche al teatro Verdi di Busseto, con una consolidata visibilità in grado di esercitare un forte richiamo internazionale. Il Festival si svolge con cadenza annuale nel periodo ottobre-novembre e comprende rappresentazioni liriche, concerti sinfonici, lirico-corali e cameristici, iniziative congressuali, attività di ricerca e formazione che coinvolgono numerose altre istituzioni pubbliche e private, tra le quali l'Istituto nazionale di studi verdiani. Con il presente disegno di legge si intende quindi proporre l'erogazione di un contributo finanziario annuo, a decorrere dal 2017, di un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Regio per l'organizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto affinché lo stesso possa svilupparsi in modo comparabile ad altri festival musicali di rilievo nazionale ed internazionale. Altrettanto nell'articolo 1 della presente legge, viene stanziato a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival. La Fondazione Romaeuropa è una delle istituzioni di maggior prestigio, in Italia e in Europa, per la promozione e la diffusione dell'arte, del teatro, della danza e della musica contemporanea. Da trentuno anni il Romaeuropa Festival rappresenta il punto di riferimento per la musica, la creazione artistica contemporanea e lo spettacolo dal vivo nella Capitale d'Italia. Il Festival Romaeuropa è nato nel 1986 all'Accademia di Francia - Villa Medici per iniziativa di Giovanni Pieraccini e Monique Veaute. Nel 2015 e 2016 ha ricevuto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. È sostenuto dalle Ambasciate di Francia e Spagna, dal Goethe-Institut e dal British Council che sono presenti, assieme a Roma Capitale e Regione Lazio, nel consiglio di amministrazione della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, che organizza il Festival. Il Festival Romaeuropa collabora inoltre

una programmazione di circa settantacinque giorni in 20 spazi della Capitale, in teatri pubblici e privati, spazi storici (come ad esempio il Palatino e le Terme di Diocleziano), musei di arte contemporanea e spazi indipendenti. Presenta una programmazione artistica internazionale di grandi maestri e sostiene il rinnovamento e le giovani generazioni italiane. Il Festival Romaeuropa collabora e produce con i maggiori festival europei, quali ad esempio Avignone, ed è membro nelle reti europee Theatron, Aerowaves, The Little Project. Nel corso degli anni Romaeuropa ha ospitato i maggiori rappresentati della musica del nostro tempo, il teatro musicale di avanguardia, la sperimentazione sonora, le nuove musiche elettroniche e le tradizioni musicali in un rapporto di incontro e dialogo con tutte le arti tra cui la danza, il teatro e le arti visive. Presenta in media oltre 40 progetti di musica e spettacolo, per circa 120 rappresentazioni, con oltre 40.000 presenze. Il Festival dedica ogni anno ampio spazio alla formazione dei giovani e del pubblico con 12 programmi e percorsi gratuiti, incontri ed approfondimenti prima e dopo gli spettacoli, ha una forte presenza sul *web* attraverso i propri canali *social*, ha un archivio storico riconosciuto dal Mibact di oltre 3.500 titoli ed è attento al rapporto tra creatività e nuove tecnologie attraverso la propria sezione Digitalife. Collabora stabilmente con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Soprintendenza Nazionale Speciale per il Colosseo e l'Area e l'Area centrale archeologica, il Teatro di Roma e l'Opera di Roma, il Macro e il Maxxi, i teatri privati della città di Roma e i centri di cultura indipendente. Crocevia di scambi culturali con il mondo intero, la *mission* del Festival consiste nell'intercettare le energie del contemporaneo per trasformarle in arte e cultura, in esperienze artistiche innovative capaci di esprimere la tensione verso il futuro e di spostare sempre più avanti la frontiera dell'indagine artistica; ma anche in nuovi modelli di sviluppo e di gestione d'impresa in ambito culturale. Fedele alla propria missione, Romaeuropa ha perseguito e raggiunto negli ultimi anni negli ultimi anni l'obiettivo di avvicinare un pubblico vasto e composito alla creazione artistica contemporanea mondiale, oltre che a promuovere la conoscenza dei grandi maestri e dei giovani talenti nel campo delle arti sceniche. *(Applausi della

rendo conto che questi argomenti importanti giungono in Assemblea quasi come scampoli rispetto a una problematica più ampia e cogente, che vede il il Paese impegnato su fronti, in alcuni casi, di vera disperazione, quali, per esempio, l'aumento della disoccupazione o la diminuzione delle assunzioni. Manca

sul Festival Verdi di Parma e Busseto tutti guardino con attenzione perché non può non dirsi utile

alla realizzazione di un più ampio e più qualificato programma, qual è, appunto, negli intenti della fondazione che sovrintende alla organizzazione di questo Festival. In questo senso, mi consenta, signora Presidente, di rivolgere un appello al Governo e alla sua maggioranza affinché possa intravedere in questa occasione, in questo dibattito parlamentare,

della manifestazione, altrettanto importante, qual è il Festival della Valle d'Itria in Puglia, forse il Festival più rilevante del Mezzogiorno dal punto di vista della qualità,

a metà degli anni Settanta, ha un padre nobile che, già con l'aver prestato il suo nome e anche la sua opera, consentito al Festival di crescere anche in termini di dignità culturale. Si chiama Paolo Grassi, l'allora sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano. Paolo Grassi, originario di Martina Franca - i genitori erano nati a Martina e poi emigrati al Nord, precisamente a Milano - volle riconoscere nella sua terra d'origine

dell'arretratezza attraverso la crescita culturale, la "inseminazione culturale". Paolo Grassi all'epoca ebbe questa intuizione, che non fu soltanto di un luminare e di un veggente dal punto di vista artistico e culturale, qual era lui, ma coinvolse anche nomi straordinari. Lo stesso Strehler ebbe la possibilità di dare a questo Festival la sua adesione morale. Pertanto, a Martina Franca ogni anno, da ben quarantadue anni, si svolge il Festival della Valle d'Itria, che fra l'altro si distingue nel panorama delle manifestazioni italiane e internazionali del genere perché ha a cuore la riscoperta dei repertori e degli autori più inconsueti della scuola napoletana e pugliese, particolarmente del Settecento e dell'Ottocento. Cito alcuni nomi: Paisiello, Piccinni, Mercadante, Traetta, Leo. Il Festival ha anche il merito di aver riportato in auge la grande tradizione operistica europea. Vanta un'affermata scuola di bel canto e ha dato vita all'artigianato di scena, producendo in proprio costumi e scenografie. Ha messo in scena in scena ben 1.500 produzioni, sin dall'anno in cui è stato fondato. Le rappresentazioni ed i concerti solitamente iniziano a metà luglio di ogni anno per chiudersi nei primi Con maggiori risorse a disposizione il Festival potrebbe allungare la stagione consentendo maggiori introiti finalizzati all'autosostentamento, generando economia per il territorio in termini di presenze turistiche già ragguardevoli per la indiscussa qualità delle produzioni artistico musicali. Per questo occorrerebbe sostenere con maggiori finanziamenti gli sforzi organizzativi della fondazione che sovrintende alla organizzazione e promozione del Festival. al Festival di raggiungere livelli organizzativi e di qualità artistica in grado di generare indotto al territorio, mettendo a sistema l'economia turistica della Murgia dei Trulli, comprensorio che raggruppa una quindicina di comunità civili dedite all'accoglienza ed alla ricettività. Soprattutto, le nuove risorse potrebbero destagionalizzare il programma artistico con indubbi benefici per i pubblici appassionati di tutto il mondo. Alla stregua di queste considerazioni reputo importante che l'Assemblea proceda all'approvazione di questo disegno di legge. Mi appello al Governo e all'Assemblea intera affinché facciano propri i *desiderata*, le ambizioni, gli sforzi, i sacrifici di una una parte del Paese, che si è spesa finora per la dignità della cultura, anche nel Mezzogiorno, affinché abbia la possibilità, non soltanto di sopravvivere, ma anche di migliorare tutto ciò, a favore dell'intera cultura nazionale e internazionale.

Qui si tratta di festival internazionali; si tratta di dare copertura stabile a dei festival che hanno un respiro internazionale. Perché il Festival Verdi non entrò nella legge n. 206 del 2012? Perché all'epoca il Festival godeva di un finanziamento speciale, legato alle celebrazioni verdiane. E fu solo per evitare una sovrapposizione di finanziamenti che il Festival, all'epoca, non

Si auspicava, cioè, che il Festival Verdi fosse inserito nel finanziamento stabile dato il respiro internazionale. Verdi è il musicista che viene più eseguito all'estero; Verdi è un ambasciatore non solo della musica italiana, ma anche della lingua italiana perché uno dei dati più rilevanti è che la penetrazione della lingua italiana passa anche attraverso i libretti d'opera, al punto tale da costringere i cantanti a diventare non degli esperti della lingua italiana, ma dei conoscitori e ad esercitarsi in un lessico che non è semplice e nella dizione. I corsi di lingua italiana per il bel canto sono attivi in tutte le parti del mondo

fare un intervento che celebri la grandezza di Verdi e l'importanza di questo finanziamento e vorrei, piuttosto, levarmi qualche sassolino dalla scarpa.

Presentammo un emendamento (che è tutto sommato lo strumento più corretto) alla legge di stabilità, perché non si trattava di istituire un principio tramite una legge, ma di integrare un finanziamento, nel pieno riconoscimento dell'importanza di queste celebrazioni. L'emendamento non venne approvato. L'emendamento era stato presentato dal senatore Pagliari, che giustamente chiese che la prima firma fosse la sua essendo un senatore del territorio.

e di un orizzonte culturale talmente ristretto da far rabbrividire: anche se lo pensi, non oseresti dirlo. L'emendamento non passò e si aprì una *querelle* con il senatore Pagliari sul territorio perché cominciò a saltare il primo milione di finanziamento fisso. Il Comune di Parma non si perse d'animo e continuò a risollevare la difficile situazione finanziaria in cui il teatro Regio ero piombato. Nessuno di noi si è perso d'animo

La legge di stabilità del 2015 ha segnato anche un altro momento curioso, perché anche allora l'emendamento fu presentato dalla sottoscritta. Non sfugge a nessuno che il sindaco di Parma sia stato sistematicamente, regolarmente, scientificamente e ripetutamente non appoggiato dal partito di cui faceva parte. Di conseguenza, visto che, nonostante il campanilismo che spesso anima i miei colleghi di oltre la Val d'Enza e visto che comunque sono di Reggio (per

che anche stamattina sui giornali viene di nuovo attaccato dalle procure. Ma c'è un giudice a Berlino e non sono tutti «cortigiani, vil razza dannata».

è stato lo strumento di educazione sentimentale, di cultura, di interesse e di aggregazione di un popolo che è molto più ampio di quello che si reca al Teatro Regio con l'abito da sera.

a Parma il Verdi Off viene sostenuto anche da una brillante e lodevole iniziativa di industriali, che si chiama «Parma, io ci sto!», con una sinergia che è quella più utile per il nostro Paese: quella che si sviluppa nei territori, che mette insieme sia la volontà e il sostegno popolari sia la capacità di coloro che hanno la disponibilità economica e che responsabilmente mettono la loro faccia su iniziative che valorizzano il territorio. Questa valorizzazione non è una marchetta, ovviamente, ma è un segno, un simbolo, un esempio: è qualcosa che va incoraggiato, va portato in giro, va seguito ed aiutato, perché può diventare un modello e un esempio da seguire.

evitare la navetta che tanto dispiace al senatore Marcucci. Senatore Marcucci, questa sgradevole navetta che vi ha spinto a modificare così radicalmente la Costituzione la possiamo evitare subito, perché nella legge di stabilità, che si sta per presentare, voi stessi potreste tranquillamente inserire questo emendamento; e se non lo metterete voi, lo faremo noi, così potremo dimostrare che ancora una volta la navetta è superabile attraverso un'azione, magari del Governo.

Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival, spero che oggi i nostri ex colleghi del Movimento 5 Stelle non riterranno che anche questa sia una marchetta.

non parliamo del festival del sindaco di Parma, bensì del Festival di una fondazione che dovrebbe essere autonoma e libera di decidere il proprio programma culturale. Se noi in quest'Aula perdiamo sempre ore ed ore a dire che i partiti e le loro segreterie devono togliere le loro mani, manine o manone dagli enti lirici, bisogna poi essere conseguenti. Quindi non perdiamoci in polemiche, che sono sempre le stesse. Credo che molti italiani che nel 2013 hanno votato quel partito oggi si siano pentiti, perché se dobbiamo trasformare ogni iniziativa legislativa in una polemica tra 5 Stelle ed ex 5 Stelle, credo sia mortificante innanzitutto per loro che, forse, credo e immagino pensassero a una stagione di cambiamento, di riforma, di proposta costruttiva e non a continui litigi che devono coinvolgere Camera e Senato anche quando trattiamo argomenti condivisi, votati tutti insieme in Commissione. Tuttavia, noi qui ricordiamo un'iniziativa lodevole, quella del Festival Verdi, che coinvolge anche la città di Busseto, proprio perché nel 2013 abbiamo anche lì sostenuto economicamente il centenario della nascita di Verdi. Voglio ricordare che il 2013 è una data importante per la lirica, perché, con un lavoro

e il rilancio dei beni culturali. All'interno di questo decreto, come ricorderanno senz'altro i membri della mia Commissione, c'era un provvedimento fondamentale, concernente i 25 milioni di euro devoluti alle fondazioni che si fossero impegnate a ristrutturare il loro debito. Voglio ricordare questo passaggio normativo importante, che ha coinvolto in modo particolare il Senato e la Commissione presieduta dall'amico Andrea Marcucci, necessario che queste 14 - un numero esorbitante - fondazioni lirico-sinfoniche abbiano un atteggiamento e un comportamento virtuosi, altrimenti il debito aumenta, non viene affatto ristrutturato e i problemi rimangono sul tappeto. A questo proposito - voglio ricordarlo soprattutto ai miei amici eletti a Roma che il Teatro dell'Opera, che pareva essere risorto grazie alla guida illuminata di Carlo Fuortes (che peraltro è anche un amico personale),

aumentati nell'ultimo anno di 10 milioni: da 44,4 a oltre 54 milioni di euro di debiti. Cosa voglio denunciare in quest'Aula? Attenzione, noi oggi approviamo -

per finanziare con un milione di euro il Festival Verdi di Parma e Busseto e il Romaeuropa Festival: due iniziative importanti, che conosco anche direttamente per averle frequentate

abbiamo il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) che destina quasi 500 milioni di euro l'anno per la cultura e le attività culturali

credo che lo Stato avesse il diritto e la responsabilità di frenare le erogazioni crescenti loro destinate. Bisogna che lo Stato possa destinare le proprie risorse a fondazioni che se lo meritano e che dimostrano

con le forze sindacali, che non possono essere, loro, padrone degli enti lirici, ma devono essere al servizio della cultura. Gli enti lirici, infatti, ricevono - lo ricordo - oltre 200 milioni di euro degli italiani, che vanno a pesare sulla fiscalità generale. I denari non nascono dall'oggi al domani: sono frutto dell'imposizione fiscale e credo che il cittadino abbia tutto il diritto di vedere gestite nel modo migliore le proprie risorse, anche dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

sono gestite in modo autorevole? La riforma Bray e, ancora prima, la riforma Bondi hanno raggiunto lo scopo oppure dobbiamo continuamente intervenire con leggi, leggine e finanziamenti? Uno infatti potrebbe anche domandarsi: come mai il Festival Verdi non era stato finanziato? E come mai poi la copertura

un'inchiesta conoscitiva su come è stato gestito in questi venti-trent'anni il Fondo unico per lo spettacolo e per il teatro, per le fondazioni lirico-sinfoniche oppure, ambiguamente e furbescamente, cominciamo con alcuni provvedimenti, come la legge sul cinema, a sganciare i vari settori della cultura dal Fondo unico? Meglio sganciarsi, quindi eliminare il FUS cinema e creare un fondo nuovo nazionale per la produzione cinematografica e per l'audiovisivo, di 400 milioni. Quindi abbiamo il "FUS 2 cinema", che noi abbiamo anche approvato; ma è necessaria trasparenza sui fondi che vengono utilizzati. Quindi, per rispondere alla senatrice Mussini, non sarà una marchetta, forse è un marchettone. Però, attenzione, qui stiamo parlando di centinaia di milioni di euro,

Cerchiamo di avviare un confronto serio anche con le forze sindacali e con tutte le associazioni di categoria, per trovare il sistema migliore per fare meglio le cose, visto che i soldi ci sono o ci sarebbero ci sarebbero e visto che sono soldi pubblici. La legge Veltroni (sempre Veltroni: fondo di garanzia per il cinema, 1.000 miliardi delle vecchie lire buttate dalla finestra per film mai fatti, mai visti, mai prodotti, mai realizzati, e tutti questi registi,

hanno tutto di pubblico (soprattutto i soldi). Ecco, vogliamo fare chiarezza su questi passaggi o vogliamo continuare con decreti, decretini e decretucci, che noi convertiamo subito, in fretta e furia, perché non possiamo dire di no alla cultura nazionale e alla nostra identità, visto che c'è sempre il centenario di turno?

la legge sullo spettacolo dal vivo, che abbiamo stralciato (perché il Governo pretendeva pure una delega) e che dovrà tornare in Parlamento. Il Parlamento allora faccia il suo dovere. Quindi, in un sussulto di dignità, cerchiamo di seguire questi passaggi, visto che la cultura, il patrimonio culturale, i beni culturali, storici, artistici, monumentali e paesaggistici sono la risorsa fondamentale e visto euro investito nella cultura produce 7 euro; cerchiamo di essere conseguenti e di fare il nostro dovere fino in fondo.

effettiva radice, dal punto di vista legislativo e anche dal punto di vista delle dinamiche di alcuni settori. Ritengo che questo provvedimento valorizzi, riconosca e amplifichi due istituzioni che, in modo diverso, fanno parte del patrimonio culturale italiano. Ovviamente, sul Festival verdiano, credo che ci siano poche parole da spendere per quanto riguarda il valore

e l'indirizzo politico del Governo e della maggioranza di mettere al centro delle politiche pubbliche la cultura come veicolo di crescita civile, d'identità e di inclusione, ma anche di ponte con altre culture.

Ciò conferma l'assoluta imparzialità della scelta della maggioranza, nel senso che, ovunque si manifesti un'istituzione degna di considerazione, questa viene finanziata a livello nazionale.

allo scontro tra Pizzarotti e altri o ritenere che il finanziamento al Festival Romaeuropa sia un riconoscimento al

disattento alle esigenze della cultura a Roma, così come lo è a quelle del resto del territorio, non essendo evidentemente priorità di questo movimento la politica in favore della cultura.

alcuni emendamenti presentati alla legge di stabilità, ancorché meritevoli di attenzione nel loro contenuto, non toglie alcunché all'interesse per quelle iniziative che la maggioranza ha avuto in ogni caso, perché - ripeto - non è la legge di stabilità lo strumento per disporre microfinanziamenti a favore di singole istituzioni.

il Festival Romaeuropa, veicolano le esperienze culturali contemporanee dei loro Paesi, facendone un luogo di conoscenza reciproca delle culture europee. La rassegna è anche diventata un luogo di aggregazione per i giovani, che trovano l'espressione della loro contemporaneità in un Festival dedicato, dedicato, nelle sue varie manifestazioni (dal teatro, alla musica, al balletto) esattamente a questo e alla contaminazione tra cultura e nuove tecnologie, che rappresenta il futuro delle espressioni culturali.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente voglio ringraziare la 7a Commissione e la relatrice per questo disegno di legge che va esattamente nella direzione auspicata dal Governo, cioè quella di

credo che le sollecitazioni dei colleghi, del senatore Liuzzi e del senatore Giro vadano considerate con molta attenzione. È vero che in Italia esistono molte iniziative meritevoli di sostegno è vero anche che esiste un problema legato all'attività ordinaria, sia musicale che teatrale, che soffre ancora per la carenza di risorse. È anche altrettanto vero che i criteri di distribuzione dei fondi pubblici devono essere oggetto di attenzione approfondita da parte di questo Ministero attraverso un nuovo decreto. nuovo decreto. Siamo perfettamente consapevoli di tutto questo e credo che in una dialettica franca e portata a sottolineare i principi di trasparenza ed efficacia, si potrà arrivare ad un risultato verso il quale sia il nostro Ministero che questo Governo vogliono puntare.

Infatti è evidente che se parliamo di ambasciatori della nostra cultura, non solo musicale, al primo posto non possiamo che trovare Giuseppe Verdi. Com'è altrettanto evidente, per quanto riguarda il Festivaleuropa, che quel Festival ha gettato un ponte verso le grandi istituzioni culturali europee fondamentali. Questa Europa affaticata e stanca, che fatica a ritrovare le proprie radici culturali e identitarie, deve poterlo fare attraverso il linguaggio della cultura. Questo è il senso del programma Europa Creativa, questo è il senso delle azioni delle istituzioni europee e penso che in questo senso noi diamo oggi anche un sostegno ad una linea che è condivisa anche da altri Paesi europei e che deve rimanere

una perequazione sociale e culturale; sollecitavamo - e sollecitiamo tuttora - una volontà da parte del Governo di intravedere anche nelle iniziative virtuose

consegnare all'attenzione di questa Assemblea gli sforzi di un'organizzazione che da quarantadue anni contribuisce a fare di quel Festival una punta di diamante di cui l'intero

alla legge Bondi, che bene ha operato e che, in effetti, adesso è riconosciuta

al Festival Romaeuropa, che è una delle manifestazioni di maggior prestigio, in Italia e in Europa, per la promozione e la diffusione dell'arte, del teatro, della danza e della musica contemporanea. Non ci Non ci dilunghiamo, in quanto condividiamo il disegno di legge e ci

un inno alla nostra lingua, alla nostra amata lingua e, da toscano, non posso che rallegrarmi di quanto è stato fatto. Signor Presidente, faccio una ultima considerazione.

È un Festival riconosciuto a livello mondiale, non solamente dagli amanti e dai fautori del Maestro, ma anche da minore. Si tratta, quindi, di un evento che non riguarda solamente, come qualcuno può pensare, la città di Parma e il territorio della Provincia di Parma, ma l'Italia intera.

che attraverso la musica e l'opera si fa politica. Era un convinto anticlericale, un convinto uomo del Risorgimento

di Parma, non mi si può certo accusare di fare una politica di natura campanilistica. Voglio riprendere una frase di Verdi: «Bandire ogni idea comunale meschina! Noi tutti dobbiamo tendere una mano fraterna, e l'Italia diventerà nuovamente la prima nazione del mondo»,

tramite l'*art bonus*. È un'attività intensa che ha a che fare con le scelte politiche sulla base di principi non sono soltanto culturali, ma anche E questa è la sede in cui parlarne. Non accetto sinceramente l'ipocrisia di chi dice: oggi parliamo di Verdi, parliamo del Maestro. Sì, oggi parliamo di Verdi, parliamo del Maestro, ma parliamo anche di un'Italia che ha bisogno di tante cose, molte di più di quelle che vengono fatte. Oggi parliamo di un Paese che, se vuole arrivare a mantenere o confermare un primato, deve fare questa come tante altre scelte che ipocritamente, invece, vengono lasciate nell'ombra. Faccio anche una precisazione, avendo la senatrice Lanzillotta

con motivazioni di natura culturali e cioè riferite alla validità di questo Festival che ha raggiunto un grande rilievo internazionale e si contraddistingue per la molteplicità delle proposte che ogni anno vengono messe in cartello. Oltre agli spettacoli sono da sottolineare gli studi e le attività di ricerca e formazione, le iniziative congressuali che coinvolgono istituzioni pubbliche e private e la ricerca di giovani talenti. Oggi possiamo anche esprimere un giudizio sul programma del Festival 2016, attualmente in corso, che presenta un calendario denso di spettacoli, concerti, incontri e giornate di studi, che si realizza in luoghi storici legati al grande musicista, quali il Teatro Regio di Parma e il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, ai quali da quest'anno e per il prossimo triennio si affianca il Teatro Farnese, un luogo di monumentale bellezza, riconquistato all'utilizzo teatrale grazie a una convenzione siglata con il Polo museale dell'Emilia-Romagna, che il Festival offre alla creatività dei grandi maestri della regia internazionale per una sfida ardua: l'allestimento di un'opera verdiana che valorizzi i limiti che la conservazione dello spazio museale impone; una vera e propria sfida che fa fare un salto di qualità al Festival anche dal punto di vista dell'innovazione. secondo intervento è a favore di Romaeuropa Festival, organizzato dalla omonima fondazione, una delle istituzioni di maggior prestigio in Italia, che propone un ricco cartellone di spettacoli i cui protagonisti sono la danza contemporanea, il teatro contemporaneo, la musica e il cinema. Ampio spazio viene riservato ai giovani che trovano una vetrina di grande importanza: l'innovazione e la sperimentazione sono la costante di tutti gli appuntamenti. Pur non essendo antichissimo - ha una trentina di edizioni alle spalle - Romaeuropa Festival è ormai riconosciuto come il più importante festival italiano in grado di presentare il meglio della creazione artistica contemporanea e vanta un pubblico di fedelissimi a cui si aggiungono ogni anno nuovi spettatori esercitando un forte richiamo anche su quelli stranieri. Entrambe le programmazioni, pur con diverse caratteristiche, hanno una rilevante connotazione internazionale e costituiscono, quindi, degli strumenti di grande importanza per divulgare la conoscenza delle località che li ospitano e per sostenere e alimentare il rilancio e la valorizzazione del nostro territorio attraverso sinergie e sforzi coordinati, con importanti ricadute positive sull'attività economica del turismo. Si afferma il principio, quindi, delle attività culturali come volano di propulsione per l'economia del nostro Paese. L'intervento finanziario a sostegno di queste due programmazioni risulta del tutto giustificato, e non lo riteniamo essere né una regalia a questo o quell'amministratore, come sembra di aver colto da alcuni interventi in fase di discussione generale. È il giusto riconoscimento e sostegno a una iniziativa di alto profilo, profilo, necessario in un periodo in cui sono più difficili gli interventi privati a favore delle iniziative culturali, e utile per dare certezza delle risorse a disposizione. A tal proposito vorrei fare la proposta - e mi rivolgo al sottosegretario Borletti Dell'Acqua - di valutare l'estensione dell'applicazione della norma dell'*art bonus* anche alle iniziative culturali oltre che al recupero di beni monumentali. Il voto di Area Popolare, come preannunciato, sarà favorevole.

nel realizzare un'iniziativa permanente che valorizzi la produzione artistica e intellettuale di un grande italiano, che è stato ed è punto di riferimento per coloro che amano il nostro Paese non soltanto per le sue caratteristiche

per due ragioni: in primo luogo, perché ho avuto il piacere di assistere personalmente a delle rappresentazioni nell'ambito del Festival Verdi e ho potuto constatare la loro qualità,

in secondo luogo, ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia che ha regalato alla lirica una delle sue voci e interpreti più apprezzate negli anni Trenta e Quaranta, e che mi ha trasmesso sin dalla tenera età interesse e amore per il bel canto, Pia Tassinari. È un buon provvedimento, questo? Sì. Poteva essere migliorato? A nostro avviso sì, ad esempio accogliendo l'emendamento, a prima firma della senatrice Blundo, che chiedeva di introdurre nella lista dei beneficiari del contributo anche il Festival Donizetti Opera di Bergamo e il Bellini Festival di Catania, nell'ottica di fare rete per meglio concertare strategie tese a valorizzare e promuovere il nostro significativo patrimonio musicale; nonché di aumentare le risorse destinate a quest'operazione. Fare rete è così importante e così difficoltoso in Italia in tanti ambiti della vita della nostra collettività. risorse: risorse esigue - a nostro avviso - che sono state assottigliate e che continuano a non essere aggiuntive; risorse che vanno ad attingere al Fondo unico per lo spettacolo, che è stato oggetto di una recente riforma, molto contestata a causa di uno scellerato algoritmo che ha sancito la chiusura e messo in pericolo la vita di tante realtà culturali;

FUS sta aspettando un provvedimento *ad hoc* da parte del Governo e del ministro Franceschini che lo rappresenta, a seguito dello stralcio dell'articolo 34 del provvedimento che disciplina il cinema e l'audiovisivo. Colgo l'occasione per osservare che il provvedimento in merito al Festival Romaeuropa e al Festival Verdi non esaurisce quanto il Governo è chiamato a fare per sanare la situazione di crisi in cui ancora versano il teatro e la danza in Italia, che ancora attendono che si traducano in concreto gli *slogan* sbandierati a più riprese. E colgo anche l'occasione per ribadire che siamo in attesa del decreto *ad hoc* che Franceschini ci ha promesso. Infine, colgo l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Assemblea

Arena di Verona. I giornali locali stanno ampiamente trattando la questione, ma poco se ne sa e si legge sui giornali nazionali di quanto sta accadendo a seguito del piano di risanamento, che vede la compromissione di molti quindi, l'attenzione del Governo e del sottosegretario Borletti Dell'Acqua, particolarmente sensibile a questi temi, affinché si metta mano in modo serio alla situazione dell'Arena di Verona e non si permettano ingerenze politiche, come è avvenuto

che dice che il Movimento 5 Stelle non è presente sui temi della cultura. Mi spiace che la senatrice Lanzillotta, così interessata alle sorti di questo provvedimento, non sia ora presente in Aula per votarlo. I suoi colleghi le ricorderanno che, se nel decreto valore cultura è stato inserito un emendamento che prevede la verifica degli interessi anatocistici corrisposti dalle fondazioni in relazioni bancarie intercorse tra le stesse e e gli istituti di credito per gli affidamenti, se questa verifica, sacrosanta e necessaria in sede di rinegoziazione del proprio debito, è stata introdotta, è stato grazie a un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle in sede d'esame del relativo

che sollecita il Governo e le istituzioni locali ad addivenire a una mappatura organica dei nostri luoghi della cultura abbandonati e in stato di degrado, per poi avviare un progetto complessivo di recupero e di destinazione programmata, attraverso programmi funzionali. È stato grazie al Movimento 5 Stelle se all'interno dell'istituzione è stato organizzato un convegno sulla archeologia industriale e sulla necessità di recuperare le aree industriali dismesse, in concomitanza con l'esame in 10a Commissione di un disegno di legge per il recupero delle aree industriali dismesse. Il Movimento 5 Stelle ha ha presentato degli emendamenti e alcuni sono molto piaciuti alla prima firmataria del disegno di legge, la senatrice del Partito Democratico Camilla Fabbri. Uno di questi emendamenti prevede il recupero di alcuni immobili, previa un'adeguata diagnosi, affinché siano destinati eventualmente a

addivenuti a una normativa che ha previsto l'istituzione di un portale e l'introduzione sistemica della pratica del *crowdfunding* e del *fundraising* in questo Paese è stato anche grazie al lavoro che il Movimento 5 Stelle ha svolto non solo in prima linea, ma anche nelle retroguardie all'interno del Ministero, per promuovere questo tipo di pratiche, confluite poi nell'*art bonus*. Quindi ditelo alla senatrice Lanzillotta. La senatrice Lanzillotta valuta il mondo guardando solo nel suo piccolo orticello di persona che non è mai stata presente in Commissione istruzione pubblica, beni culturali

La legge n. 196 del 2009 prevede l'esclusione per legge degli interventi microsettoriali. Tutti dovrebbero essere resi inammissibili, perché la legge di bilancio è programmatica e, quindi, in quella sede casomai bisognava prevedere un fondo unico da destinare a tutti i festival e demandare poi a una gestione successiva la programmazione dei fondi, perché il rischio - come succede in questa legge - è che forse i fondi si potranno rivelare insufficienti. Nonostante questo per tutte le ragioni che ho elencato il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo disegno di legge, perché non si dica che il Movimento 5 Stelle utilizza i disegni di legge a fini politici e perché si dica che il Movimento 5 Stelle

È iscritto a parlare il senatore Giro. Ne ha facoltà.

un passaggio legislativo importante, avendo votato in quest'Aula pochi giorni fa lo stralcio della delega affidata al Governo sullo spettacolo dal vivo. Quindi, cerchiamo di fare - come ho detto in precedenza - il nostro dovere fino in fondo cerchiamo soprattutto di spalancare finalmente una volta per tutte le porte di questo importante settore della cultura nazionale, che noi vantiamo in tutto il mondo e che il mondo ci invidia,

sull'importo donato per la riqualificazione del patrimonio culturale. Possiamo moltiplicare le iniziative finalizzate a sostenere un settore che è in crisi - come abbiamo visto - e che è oberato da debiti milionari, dando una possibilità al privato. Ma il privato interviene se ci sono un quadro e un sistema chiaro di rapporti di reciproca lealtà, dove si sa chi fa cosa e non dove si chiede e si pretende soltanto, mentre il privato si deve limitare a erogare in modo univoco, senza partecipare alla costruzione di un progetto. Ho sempre in mente la vicenda paradossale di Diego Della Valle che, dopo molte traversie giudiziarie, è dare allo Stato 25, 30 milioni di euro per il restauro integrale del Colosseo, un monumento straordinario, forse il più visitato in Italia.

cogliere l'opportunità di riscrivere una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi in modo condiviso, coinvolgendo le Commissioni di merito di Camera e Senato, che hanno al riguardo ancora molto da dire e

so bene che questo riconoscimento comporta una missione cui noi parmigiani cercheremo di dare seguito. Voglio ringraziare la Commissione cultura e il Presidente del Gruppo;